Così come è stato deciso, ogni anno è necessario che la Commissione riferisca all'Aula

tali che producessero non elementi di carattere casuale o occasionale, ma elementi capaci di fornire un quadro esatto e quanto più compiuto del problema

trasporti ed infortuni *in itinere* (coordinato dal senatore Morra); formazione e prevenzione (coordinato dalla senatrice Bugnano); verifica dello stato di attuazione della nuova normativa di cui alla legge n. 123 del 2007 e al decreto legislativo n. 81 del 2008,

nostro lavoro abbiamo cercato di coinvolgere tutti i componenti della Commissione a studi più approfonditi e a conoscenze più mirate per poter dare le risposte a cui prima ho fatto cenno.

proprio da alcuni passaggi di queste audizioni per dare il taglio del metodo di lavoro che si è seguito.

compresa l'elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Non posso non far presente la problematicità, che anche i sindacati dei lavoratori hanno esternato,

e richiede un'attenzione sempre maggiore per fare in modo che incidenti ed infortuni, anche mortali (moltissimi dei quali accadono proprio nelle piccole imprese) possano essere prevenuti.

del coordinamento e della sinergia tra i diversi soggetti istituzionali competenti, sia a livello centrale che periferico. In particolare, posto

Credo si debba serenamente riflettere sull'esigenza di superare il conflitto o l'incomprensione che talvolta si determina

dell'appostazione di bilancio del piano sanitario nazionale 2006-2008 relativa alla prevenzione potesse essere definito in riferimento alla prevenzione degli infortuni e delle malattie, quindi della salute nei luoghi di lavoro. Purtroppo come Commissione non riuscimmo ad ottenere un impegno da parte del rappresentanze della Conferenza Stato-Regioni (e certo non per colpa di quel rappresentante, stimatissimo, della Regione Toscana,

nel senso che le Regioni avrebbero comunque svolto un certo numero di attività di prevenzione e di controllo. penso che lo Stato debba ricoprire un ruolo di indicazione esclusivo per quanto riguarda il tema della prevenzione degli infortuni e della salute nei luoghi di lavoro,

al sistema di protezione tedesco contro il rischio di infortuni sul lavoro, segnalo che in Germania la potestà legislativa in materia di sicurezza e salute del lavoro spetta in via esclusiva allo Stato.

la potestà legislativa in materia di sicurezza e di salute sul lavoro spetta in via esclusiva allo Stato centrale, che emana norme valide su tutto il territorio nazionale, tenendo conto anche delle direttive comunitarie in materia. I singoli Länder possono emanare norme di dettaglio, ma non derogare alle leggi federali, delle quali curano l'applicazione a livello locale e, insieme alle casse assicurative professionali, i relativi controlli. Un ruolo importante nel processo legislativo e regolamentare del settore è svolto anche delle parti sociali, che elaborano di comune accordo linee guida per i loro aderenti o proposte normative, sottoposte al vaglio e all'approvazione dello Stato. A livello centrale, competente per il settore degli infortuni sul lavoro è il Ministero federale per il lavoro e la sicurezza sociale, che ha il compito di promuovere un lavoro di qualità all'interno delle imprese e di creare le condizioni ambientali adatte ad un lavoro sicuro. Accanto alla normativa sulla tutela e la prevenzione del rischio, in questa legislatura in Germania sono stati finanziati programmi per migliorare la vivibilità all'interno delle aziende e sui luoghi di lavoro, con la partecipazione degli enti locali e delle parti sociali.

in questa rete di protezione anche gli enti locali, perché sono le realtà in cui in modo più specifico si conoscono e si analizzano elementi che possono condizionare problemi di pericolosità e di rischio, non solo in riferimento a possibili infortuni e quindi al diretto coinvolgimento del lavoratore, ma anche a danni che potrebbero arrecarsi all'ambiente. Desidero ricordare,

e al contrasto degli infortuni, ma anche le problematiche più ampie di contesto del territorio. Mi sembra che questo ragionamento possa sicuramente essere colto, anche perché da più parti ci viene detto che i sindaci gli amministratori locali non hanno alcun elemento di informativa su taluni problemi che comunque riguardano il loro territorio. In Germania - lo dico per conoscenza e

In Francia, il sistema di protezione contro il rischio di infortuni sul lavoro ha un'articolazione alquanto complessa e, comunque, la competenza legislativa appartiene allo Stato centrale;

Nell'ambito del Governo, le competenze in materia di sicurezza e salute del lavoro fanno capo a più dicasteri; al Ministero del lavoro, delle relazioni sociali, della famiglia e della solidarietà, attraverso la Direzione generale del lavoro, per quanto concerne gli aspetti della prevenzione e dei controlli; al Ministero della salute, della gioventù e degli sport e al Ministero del bilancio, dei conti pubblici e della funzione pubblica, attraverso la Direzione

di sicurezza sanitaria dell'ambiente e del lavoro (AFSSET) che ha funzioni di consulenza scientifica e di sostegno alla ricerca». Credo che noi, anche da questo punto di vista, dovremmo rivedere e rafforzare l'attività perché in effetti è uno strumento scientifico di ricerca di altissime professionalità, che credo debbano essere da noi guardate con attenzione. Signor ci sono dei tempi dandovi qualche elemento ancora sul Regno Unito. Anche in questo Paese, la competenza legislativa in tema di salute e sicurezza del lavoro appartiene allo Stato centrale, attraverso il Ministero del lavoro e delle pensioni. del lavoro e delle pensioni. Questa attività si svolge in stretto coordinamento con le autorità locali, con le parti sociali e con i componenti del settore pubblico e privato. e privato. I colleghi che vorranno avere maggiori elementi li troveranno nella relazione pubblicata; mi corre l'obbligo però di

Questa attività si è sempre esplicata mediante uno stretto e costante raccordo istituzionale con il Governo e le Commissioni parlamentari competenti in materia. materia. Dobbiamo ricordare in modo particolare la discussione al Senato del disegno di legge n. 1305, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. Nel corso dell'esame in Assemblea, era stata presentatA una serie di emendamenti che riguardavano il decreto legislativo n.

in modo particolare sugli articoli 2-*bis* e 15-*bis* dove, a nostro avviso, si rilevavano elementi critici soprattutto nell'identificazione delle responsabilità del datore di lavoro

11a Commissione, ha recepito quanto da noi evidenziato. Lo stesso ministro Sacconi si è mostrato immediatamente disponibile a farlo e credo che abbiamo contributo anche ad evitare talune distorsioni. Mi auguro che la Commissione possa continuare a svolgere con serenità il proprio lavoro e che, così com'è stata approvata all'unanimità questa relazione

La discussione che ci accingiamo ad avviare ha al centro la necessità di tutelare la garanzia dei lavoratori a svolgere le proprie mansioni in un ambiente più sicuro. La sicurezza sui luoghi di lavoro è un diritto irrinunciabile e diventa condizione necessaria per lo svolgimento di qualsiasi attività. Quasi ogni giorno in Italia, dal Nord al Sud del Paese, siamo costretti a registrare incidenti sul lavoro, spesso causati dal mancato rispetto dei parametri di sicurezza; quindi, questo dato ci impone di dare priorità e attenzione assoluta a questo problema attraverso l'incentivazione e il sostegno ad attività che promuovano la diffusione delle norme e degli strumenti di prevenzione.

per cogliere lo spirito di collaborazione fattiva che ha animato i commissari della maggioranza e dell'opposizione. Abbiamo incontrato rappresentanti dei sindacati ed esponenti del mondo imprenditoriale, svolto audizioni, missioni in Italia e all'estero e ci siamo avvalsi dell'opera di consulenti, animati dalla convinzione che su questioni che riguardano prima di tutto la civiltà di un Paese e la tutela dei lavoratori è una di queste - non si può e non si deve discutere per far prevalere ragioni di parte. Il concetto di tutela del lavoratore va esteso in senso più ampio anche alla protezione della famiglia, dal momento che un incidente, e ancor più una vittima sul lavoro, è un evento tragico che coinvolge più di una persona, dal punto di vista psicologico ma anche materiale; per questo siamo tenuti ad andare oltre l'aspetto emotivo e ad inserire la norma disponendo, per quanto in nostro potere, che essa venga rispettata con precise garanzie. Nell'auspicio che il Governo faccia la sua parte valorizzando l'iniziativa della Commissione e provvedendo a stanziare le risorse necessarie a tradurre in fatti le disposizioni della legge, non a caso,

promuovere le iniziative opportune, con finanziamenti adeguati, per assicurare tutte le condizioni di sicurezza sui luoghi di lavoro a tutela dei lavoratori per ridurre ogni tipo di infortunio, nonché le malattie professionali attraverso controlli rigorosi e attività di prevenzione; formazione e l'informazione dei lavoratori, mettendo in cantiere consistenti forme di sostegno, in particolare alle piccole e medie imprese, prevedendo speciali premialità per quelle più efficienti su questo fronte; intervenire con un piano di verifica per assicurare salubrità e sicurezza a tutti i luoghi di lavoro di proprietà pubblica. Da assessore regionale della Campania ai lavori pubblici, ho disposto l'inserimento nella legge regionale sugli appalti, sulle forniture e sui servizi la clausola degli incentivi per le imprese attente al potenziamento della sicurezza sui luoghi di lavoro. La sicurezza va potenziata spingendo anche sulla leva della formazione dei lavoratori e dirigenti, dell'informazione con campagne mirate, ma bisogna insistere pure sui controlli e, qualora si riscontrino carenze, occorre sanzionare. A tal fine è auspicabile un coordinamento più stretto tra tutti i soggetti deputati alle verifiche: bisogna superare la logica dei controlli a campione ed operare uno sforzo più spinto per stringere la maglia della vigilanza. Quindi, occorrono molti più controlli. Ancora, resto profondamente convinto della necessità di una regolamentazione più severa che disciplini l'accesso di quanti intendono lavorare da imprenditori, per esempio nel settore dell'edilizia.

Anche avvalendoci della consulenza di istituti quali l'ISPESL (Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro), e delle dichiarazioni raccolte in audizione dei rappresentanti delle associazioni datoriali e sindacali del settore, edili), riteniamo vada segnalata come prioritaria l'esigenza di incrementare la formazione obbligatoria per tutti i nuovi assunti su cantieri edili, per cui probabilmente non bastano le 16 ore di formazione, ma bisogna farne di più. Un'altra proposta dell'ANCE, che insieme al CNR, al Ministero del lavoro, all'INAIL, all'ISPESL e a tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione deve lavorare per rivisitare il Testo unico sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, è l'utilizzo, mediante il progetto «Cantiere intelligente», di sistemi tecnologici, quali sensori, per segnalare il mancato rispetto della sicurezza sui cantieri. Ancora, abbiamo concentrato la nostra attenzione sulla necessità di controllare e sottoporre a verifiche periodiche le cosiddette opere provvisionali, ossia ponteggi, strutture e attrezzature da lavoro, noleggiate dalle imprese per allestire i cantieri. A tal proposito, nella relazione sono state proposte modifiche al cosiddetto Testo unico per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, come per esempio l'introduzione dell'obbligo per chiunque venda, noleggi o conceda in locazione opere provvisionali di attestarne l'idoneità e la previsione di incentivi per la rottamazione di attrezzature obsolete. Altra priorità riguarda i piani per la sicurezza, da redigere con maggiore attenzione, dal momento che, nonostante le tragedie che continuano a verificarsi sui cantieri - ma vale anche per gli altri luoghi di lavoro - esistono piani di sicurezza scritti male, con costi spesso sottostimati o addirittura non evidenziati. Vorrei richiamare la vostra attenzione su un ultimo punto che riteniamo - mi sia consentito il gioco di parole - di importanza vitale. La sicurezza dei lavoratori e dei cittadini non può essere ridotta a voce di spesa da abbattere, come purtroppo accade nel nostro Paese, specie nelle zone a più alta densità criminale. E allora bisogna eliminare il massimo ribasso d'asta. In questo senso, ci auguriamo che il Governo intervenga presso l'Unione europea affinché si riveda la direttiva sul massimo di ribasso d'asta per l'offerta più vantaggiosa per gli appalti pubblici. È necessario fissare un limite perché, soprattutto in alcune zone del Paese, come il Sud, ribassi ribassi d'asta eccessivi e, in molti casi, subappalti comportano il rischio di infiltrazioni malavitose e spesso si traducono in carenza di garanzie per la sicurezza sui cantieri.

oppure rimanda ad inquietanti anomalie che devono farci interrogare sulla provenienza delle risorse finanziarie cui accedono quelle ditte. Che sia l'uno o l'altro caso, non possiamo restare a guardare. Anche per questo, nel nostro Paese si continua a morire per lavoro. Ciò è inaccettabile. Vi è pertanto la necessità di agire nel concreto per segnare un cambio di passo ormai non più rinviabile in un Paese che voglia dirsi civile. auspico, a nome del Gruppo del PD, che, alla fine, si possa pervenire ad una risoluzione unitaria, come, ad esempio, la relazione di indirizzo dibattuta all'interno della Commissione monocamerale.

che fa riferimento alla civiltà di un Paese, un indirizzo univoco per attuare il decreto n. 81 nel tentativo di eliminare tragedie che sono il segno di una mancanza di attenzione e di civiltà da parte degli organi istituzionali. In merito, non possiamo che dare una risposta in termini di condivisione e di responsabilità ampia e diffusa di tutto il Parlamento. Signor Presidente del Senato, signori senatori, signori del Governo, c'è un aspetto degli infortuni sul lavoro che viene sempre molto poco, se non addirittura per nulla, considerato. riferisco ad una categoria di lavoratori ed ex lavoratori negletta e particolarmente trascurata: i lavoratori colpiti da malattie professionali, in particolare da sostanze cancerogene e genotossiche o fibre*killer* come l'amianto, che in Italia sono molti di più di quanti comunemente si creda. Nelle ordinarie ‑ per così dire ‑ statistiche sugli infortuni sul lavoro essi non sono fatti rientrare, forse perché, in caso contrario, i numeri ed i dati balzerebbero bruscamente in alto e colpirebbero in maniera troppo evidente la sensibilità dell'opinione pubblica. vengono trascurati nonostante ormai, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, le malattie professionali siano equiparate agli infortuni sul lavoro anche ai fini giuridici, sia penali che civili. almeno a tre volte tanto all'anno le vittime delle malattie professionali rispetto a quelle degli infortuni traumatici sul lavoro: vittime colpite in maniera ancora più subdola e drammatica a causa del lungo decorso del tempo

Queste non sono considerazioni astratte, ma conclusioni tratte dal contatto quotidiano con lavoratori ex esposti all'amianto, pesantemente ostacolati e presi in giro dalla burocrazia. E quando ci sarebbe bisogno di una nuova normativa, a tutela ad esempio degli ex esposti all'amianto, Parlamento e Governo da anni non rispondono; ancora oggi, con i ritardi della Commissione lavoro nell'esame dei disegni di legge in materia di amianto, si nascondono da anni dietro la necessità di verifiche e difficoltà finanziarie: continuano a lasciar morire lavoratori e cittadini inermi colpiti dalla fibra *killer*. Tra qualche settimana, la prima di novembre, si terrà a Torino la seconda Conferenza nazionale sull'amianto dal titolo: "Amianto e giustizia"; meglio sarebbe stata titolarla: "Amianto e ingiustizia".

la pervicacia e l'ottusa mancanza di volontà di questo Governo e del Ministro del lavoro e della salute a dare seguito al fondo per la tutela delle vittime dell'amianto, già istituito con l'ultima legge finanziaria 2008 del Governo Prodi e già finanziato (mentre il Governo Berlusconi ed il ministro Sacconi nemmeno rispondono alle nostre ripetute interrogazioni e sollecitazioni volte alla urgente emanazione del regolamento necessario a far funzionare il fondo, per la cui emanazione è scaduto il termine previsto dalla legge da oltre un anno: e le vittime aspettano). In terzo luogo, registreremo ancora una volta le resistenze, le negligenze, la riottosità, i comportamenti vergognosi di enti previdenziali ed assistenziali che continuano ad usare e ad interpretare la legge contro i lavoratori con comportamenti dilatori e defatigatori. luogo, registreremo le carenze di una sorveglianza sanitaria assolutamente inefficiente e diseguale sul territorio nazionale. Non è un caso probabilmente che succeda tutto questo, se consideriamo come il Ministro del lavoro stia mantenendo la sua promessa elettorale di ridurre controlli e verifiche reali ed efficaci per rispetto di tutta la normativa sulla sicurezza nel lavoro, con l'intenzione di ridurre le sanzioni. Promessa, quella del Ministro, di sollevare le imprese da doveri costituzionali sulla sicurezza che sarebbero intangibili, e accompagnata dal tentativo di introdurre nuove norme salva manager. Nei confronti di tutti i lavoratori colpiti, in particolare, da amianto, lo Stato ha da decenni un obbligo morale, etico, sociale e politico di intervenire, perché per anni, pur conoscendo la natura cancerogena delle sostanze e dei materiali trattati, ne ha autorizzato la lavorazione e la diffusione, ha omesso di intervenire, come imposto dalla scienza e dalla normativa europea, con ciò determinando le condizioni per l'insorgere e il diffondersi di malattie professionali, morti, inquinamento dei nostri territori,

che c'è ancora tempo, signori del Governo, per intervenire. Intanto, però, ricordatevi che le morti a causa dell'amianto e degli infortuni sul lavoro non aspettano la vostra negligenza, la vostra indolenza, il vostro disinteresse.

Nell'ambito della Commissione di inchiesta sugli infortuni sul lavoro ho avuto l'opportunità - avevo dato la mia disponibilità e ringrazio il Presidente e i colleghi per avermelo permesso - di

rispetto a quei datori di lavoro che non investono nell'ambito della materia antinfortunistica e che non tengono comportamenti adeguati, diretti o indiretti, a tutela dei lavoratori.

all'importanza della formazione dei datori di lavoro e dei lavoratori, soprattutto per quanto riguarda le piccole e le medie imprese;

la propria carenza in questo settore e denuncia esso stesso situazioni in cui non sempre il datore di lavoro - penso, per esempio, al mondo degli artigiani - è sufficientemente a conoscenza, sufficientemente formato in questo campo. Però questo mondo, essendo consapevole

che devono svolgere all'interno delle aziende. Vi sono poi settori (penso per esempio al settore dell'edilizia,

dell'edilizia, in cui sono importantissimi l'aggiornamento e la crescita delle competenze professionali degli operatori dei servizi, una crescita che deve svilupparsi svilupparsi anche orientando il personale verso quelle che dagli stessi operatori sono definite le buone pratiche. Sul discorso delle buone pratiche, nelle audizioni che sono state svolte nel gruppo di lavoro formazione e prevenzione (penso ai rappresentanti della Direzione generale per le attività ispettive del Ministero del lavoro, penso ad alcuni rappresentanti dei coordinamenti tecnici della Conferenza Stato-Regioni o ai rappresentanti della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione), da tutte le parti, quindi dagli operatori del settore, è stata evidenziata l'importanza delle buone pratiche e l'importanza della condivisione delle stesse. La formazione è ovviamente finalizzata al cambiamento dei comportamenti da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori, perché sappiamo che la normativa non sempre viene rigorosamente applicata. Quindi spesso capita che, anche in assoluta buona fede, non si rispettino quelle norme minime di tutela che molte volte sarebbero sufficienti a salvare la vita di un lavoratore.

aiutare i colleghi che non hanno ancora avuto modo di leggere la relazione per la discussione che seguirà), vi sono la necessità - come ho già detto - di investire maggiori risorse nella formazione e prevenzione; una verifica dell'efficacia delle attività che sono state realizzate dalle Regioni in forza di un protocollo d'intesa fra il Governo e le Regioni; la necessità di favorire una crescita nelle professionalità del personale ispettivo e delle ASL; (l'ho già detto, ma lo ripeto) di fare formazione ai lavoratori e ai datori di lavoro; infine, la necessità di realizzare una cosa che forse può apparire banale, ma che da tutte le parti è stata invece indicata come un elemento di vitale importanza, che dovrebbe far parte di quei decreti attuativi che nella nostra risoluzione vengono sollecitati al Governo, ossia l'istituzione del cosiddetto libretto formativo. Dicevo che potrebbe apparire una banalità ma ci è stato evidenziato da tutti gli operatori del settore essere, potenzialmente, uno strumento utilissimo per quanto riguarda la formazione e la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

svolto in modo unitario e con senso di responsabilità. Ritengo, però, che la relazione che avete avuto modo di leggere o che leggerete sia solo un punto di partenza. Sono ancora molte le cose da fare e auspico anch'io che si possa arrivare in quest'Aula a una risoluzione unitaria, proprio perché l'importanza e l'attenzione in modo trasversale su un tema come quello degli infortuni sul lavoro devono devono portarci a superare le contrapposizioni politiche che su altri temi possono esservi, poiché tutti dobbiamo avere lo stesso tipo di interesse per arrivare

Signor Presidente, principalmente vorrei porgere il mio ringraziamento a tutti i componenti della Commissione per il lavoro svolto, e soprattutto al presidente Tofani, che

importante e molto delicata nell'ambito della nostra società e del nostro vivere civile. Nel mio intervento vorrei soffermarmi su due aspetti trattati nella Commissione e riportati anche nella relazione intermedia,

Per quanto riguarda l'attività di vigilanza, la Commissione ha avuto modo di verificare nel corso della sua inchiesta l'esigenza di rafforzare, in maniera sempre più incisiva, il coordinamento e la collaborazione fra tutti gli enti istituzionali che si occupano, a vario titolo, della tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, sia a livello centrale che locale, secondo quanto espressamente previsto dal Testo unico. In taluni casi, infatti, in questo campo si rileva ancora una sovrapposizione e una duplicazione di competenze (ad esempio nella fase ispettiva e di controllo) che certamente non aiuta l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa. Si tratta in verità di un problema annoso, che si ricollega, da un lato, a quello più generale di razionalizzazione degli enti previdenziali ed assistenziali e, dall'altro, a quello del complessivo rapporto tra Stato e regioni nelle materie di legislazione concorrente. Tali questioni sono entrambe da tempo all'attenzione della riflessione politica su questo fronte ma sono, evidentemente, temi assai complessi, la cui soluzione definitiva richiederà ancora del tempo. Si potrebbe comunque lavorare immediatamente all'elaborazione di procedure standardizzate per la redazione di linee guida finalizzate alla stesura dei verbali ispettivi utilizzabili dagli organi preposti, al fine di promuovere l'uniformità della normativa vigente. Ricordo che oggi gli organi ispettivi di vigilanza dispongono di modelli in bianco da compilare in maniera discrezionale nell'ambito dell'ispezione nei luoghi di lavoro. La pianificazione dei modelli standardizzati per la stesura di verbali ispettivi adottabili dagli organi competenti garantirebbe, quindi, anche una migliore efficacia nell'ambito del sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi del lavoro, prevista dall'articolo 8 del Testo unico. Tale ruolo, cioè l'elaborazione delle procedure standardizzate di cui parlavo, dovrebbe essere affidato alla Commissione consultiva di cui all'articolo 6 del decreto n. 81 del 2008, di concerto con il Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui all'articolo 5 dello Il secondo aspetto su cui vorrei soffermarmi riguarda il comparto dell'istruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Qui si rilevano due problemi fondamentali: in primo luogo, la formazione. la formazione. La Commissione ha ribadito la propria profonda convinzione della necessità di promuovere la più ampia diffusione della cultura della sicurezza all'interno della scuola, come passo indispensabile per una più efficace opera di prevenzione contro gli infortuni e le malattie professionali. L'articolo 11 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del resto, già prevede la possibilità di attivare specifici percorsi formativi su tali tematiche all'interno delle scuole, sia pure nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. Ci risulta che attività formative del tipo indicato siano state avviate in alcuni istituti scolastici, in via sperimentale. Proprio al fine di approfondire la questione e dare nuovo impulso a questa importante iniziativa, la Commissione intende intensificare la propria collaborazione con il Dicastero di settore.

in maniera esaustiva per quanto concerne l'assolvimento dei propri obblighi in materia di salute e sicurezza. Faccio riferimento ai corsi di formazione per i responsabili dei lavoratori per la sicurezza (gli RLS), per i dirigenti, i preposti, gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione per gli addetti ai servizi antincendio e primo soccorso. Inoltre, il Ministero dovrebbe contribuire ad un chiarimento definitivo in merito agli obblighi di applicazione della medicina del lavoro

siano spesso ospitati in edifici o strutture obsolete, che avrebbero bisogno di importanti e purtroppo costosi interventi di adeguamento. I dati negativi in merito allo stato di carenza degli edifici scolastici, sia dal punto di vista strutturale che della mancanza di certificazioni certificazioni (statiche, antincendio o di adeguamento degli impianti elettrici), ormai li conosciamo tutti ed è superfluo ribadirli in questo consesso.

di azioni da intraprendere debba prevedere i seguenti capisaldi: una programmazione immediata degli interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici,

attivazione della normativa inerente il fascicolo del fabbricato per gli edifici scolastici e la costituzione della banca dati delle certificazioni dei medesimi edifici; verifica della ricettività degli edifici scolastici e razionalizzazione dei processi funzionali e degli spazi disponibili. Inoltre, bisognerebbe promuovere sia incisive iniziative di raccordo, coordinamento e cooperazione tra le istituzioni scolastiche ed educative e gli enti locali, finalizzate agli scambi di informazioni, alla programmazione e alla gestione degli interventi di cui ai punti precedenti, sia protocolli di gestione e relative assunzioni di reciproche responsabilità tra gli enti proprietari degli edifici scolastici (Comuni e Province) e istituzioni scolastiche,

Tale decreto dovrà affrontare anche il coordinamento e rivedere eventualmente le competenze e gli obblighi riguardanti i dirigenti scolastici e i titolari degli edifici scolastici.

il Presidente ed i componenti della Commissione per il lavoro svolto: un lavoro certosino, accurato, fatto di audizioni e sopralluoghi, sia all'estero che in Italia. Abbiamo ascoltato gli enti istituzionali preposti alla prevenzione ed al contrasto degli incidenti sul lavoro (INAIL, IPSEMA, ISPELS) e quelli investiti della funzione di di enti erogatori di prestazioni ed indennità collegate ad una menomazione e/o disabilità riconducibile ad una causa di servizio (INPS, INPDAP). Abbiamo aperto un dialogo costante con i soggetti coinvolti nel fenomeno degli infortuni sul lavoro: le organizzazioni sindacali, quelle datoriali di lavoro e dei lavoratori, quelle imprenditoriali, gli esperti della sicurezza, quali medici del lavoro, ingegneri, specialisti in prevenzione ed igiene del lavoro. Ciascuno, per la parte di propria competenza, ha evidenziato le criticità e le problematiche derivanti dall'applicazione del Testo unico. Ad esempio, i rappresentanti del mondo imprenditoriale hanno biasimato i troppi adempimenti formali e burocratici e l'inasprimento dell'apparato sanzionatorio. Come dare loro torto? Noi della Lega Nord abbiamo sempre creduto che una reale tutela dei lavoratori sui luoghi di lavoro ed una concreta conoscenza dei rischi di incidenti sul lavoro si perseguano ispirandosi ad una logica di prevenzione, informazione e formazione continua, sia sul campo che in Aula, che tenga conto delle dimensioni aziendali e delle specifiche esigenze dei diversi settori produttivi: una prevenzione mirata, accompagnata, sì, da adempimenti formali e misure sanzionatorie, ma con una correlazione alla maggiore rischiosità. L'ultimo rapporto INAIL sugli infortuni sul lavoro relativo all'anno 2008 ha confermato che, come per gli anni precedenti, i settori con indice di frequenza infortunistica di gran lunga più elevato sono la lavorazione dei metalli (siderurgia, metallurgia), la lavorazione dei minerali non metalliferi (materiali per edilizia, vetro, ceramica), la lavorazione del legno e le costruzioni, evidenziando che la maggiore rischiosità si registra nelle aziende con oltre 30 dipendenti. Sempre secondo il rapporto, i decessi per infortuni sul lavoro sono passati da 1.207 nel 2007 a 1.120 nel 2008, dato questo confortante in termini relativi, se si pensa che - come lo stesso Istituto ci ha riferito - dal 1951 è il primo anno che il numero degli infortuni mortali è sceso al di sotto dei 1.200 casi l'anno; scoraggiante, invero, in termini assoluti perché è impensabile al giorno d'oggi morire di lavoro: le cosiddette morti bianche non sono e non devono divenire un malessere della nostra società; piuttosto, devono rappresentare episodi sporadici, tesi a scomparire nel tempo definitivamente. Peraltro, gli stessi dati ci dicono che oltre la metà degli infortuni sul lavoro è da ricondursi ad errori di procedura ed a condotte soggettivamente inadeguate più che a carenze strutturali degli ambienti di lavoro. Per questo, riteniamo fondamentale procedere anche in una capillare opera di sensibilizzazione e di diffusione di una cultura antinfortunistica, a cominciare dall'età scolare. Ben venga, dunque, il dibattito in quest'Aula sul lavoro svolto dalla Commissione d'inchiesta, che rappresenta per noi l'occasione per far comprendere la drammaticità delle questioni che abbiamo affrontato, e che continueremo ad affrontare, per richiamare l'attenzione dell'Esecutivo su talune importanti questioni inerenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, sui quali la politica si è impegnata a dare risposte certe.

Probabilmente per motivi di tempo, nella relazione del senatore Tofani non si è affrontato tale aspetto, ma studiando la relazione in effetti si fa menzione del numero crescente di lavoratori non italiani che sono non soltanto regolarmente impiegati, ma anche regolarmente iscritti agli istituti

Si è più volte auspicato di pervenire ad un testo ampiamente condiviso sulla materia e anch'io sono favorevole a che si trovi una soluzione di consenso. Credo però che, oltre a trovarci d'accordo su alcune

la riforma della nostra legislazione in materia di lavoro e, dall'altra (e qui torno al centro del mio intervento), il modo con cui negli ultimi 18 mesi si è affrontata la presenza sul suolo nazionale di non italiani debbano essere radicalmente rivisti. Si dice nella relazione che «un'attenzione particolare si è sviluppata negli ultimi anni per gli infortuni ai lavoratori stranieri, le cui iscrizioni all'INAIL nel 2008 hanno superato quota 3.266.000:

di infortunio o comunque di possibile infortunio. A Caserta, secondo i dati forniti alla Commissione in occasione del sopralluogo, nei primi nove mesi del 2008 si sono riscontrati in provincia 3.202 infortuni sul lavoro, pari al 15 per cento dei quasi 23.000 casi registrati in tutta la regione Campania, con un leggero calo rispetto al 2007, quando si sono avuti 3.431 incidenti. I comparti sono sempre gli stessi: in particolare l'edilizia, ma anche l'agricoltura in quella zona. Perché mi soffermo su Caserta? Forse alcuni senatori sapranno che sabato scorso si è tenuta a Roma una grande manifestazione antirazzista, con quasi 200.000 persone che pacificamente hanno partecipato ad una marcia che si è snodata per le vie

e cioè di riprendere in considerazione la possibilità di ampliare la regolamentazione di chi oggi si trova in Italia ad altre professioni che non siano la colf o la badante. evince infatti chiaramente dai dati contenuti in questa relazione che sono tantissimi i lavoratori oggi presenti in Italia che svolgono lavori extradomestici nei campi, nelle fabbriche o nei cantieri, fino ad arrivare ai ristoranti e a tutte le varie mansioni. Se si inizia ad intravedere una soluzione condivisa relativamente al problema degli incidenti sul lavoro, ci dobbiamo porre allo stesso tempo il problema di chi non ha diritti in questo Paese, pur lavorando, e ha necessità di vedere comunque rispettati

in Italia. Il rispetto della legalità è quanto ci hanno chiesto le 3.000 persone rimaste 48 ore in più a Roma, quasi tutte provenienti dal Ghana, dalla Nigeria, dal Senegal e dalla Costa d'Avorio. Ci siamo impegnati, se non altro, a portare la loro voce all'interno del Parlamento

Signor Presidente, come Italia dei Valori non siamo mai stati entusiasti di fronte all'istituzione di Commissioni parlamentari che hanno costi elevati e tempi lunghi. Tuttavia, di fronte all'emergenza degli incidenti sul lavoro, pensavamo - e lo pensiamo tuttora - che questo fosse l'unico strumento percorribile per delineare un quadro completo e stabilire gli interventi legislativi necessari. Considerazioni oggi ancora più valide, soprattutto alla luce del decreto correttivo del Testo unico sulla sicurezza, che ha fatto di un buon testo sulla sicurezza sul lavoro una legge incerta e incompleta, sottoposta a tagli e modifiche, e di cui ancora non sono stati emanati i decreti attuativi. Il fenomeno delle cosiddette morti bianche ha assunto negli ultimi tempi proporzioni devastanti: ogni anno in Italia, da Nord a Sud, migliaia di persone perdono la vita per incidenti causati dalla mancata messa in sicurezza dei luoghi e degli strumenti su cui stanno esercitando il proprio lavoro. Secondo le stime ufficiali dell'INAIL gli infortuni denunciati nel 2008 sono circa il 4,1 per cento in meno rispetto all'anno precedente. Effettivamente, negli ultimi otto anni l'INAIL ha registrato un *trend* decrescente, ma dobbiamo anche tener conto del fatto che in quelle stime sono completamente assenti i lavoratori in nero, fenomeno che per ovvie ragioni si sviluppa soprattutto in contesti produttivi di piccole dimensioni e che investe, per altrettanto ovvi motivi, la manodopera straniera e clandestina. Immigrati clandestini sfruttati, caporalato, datori di lavoro senza scrupoli che utilizzano manodopera straniera e clandestina in condizioni di rischio elevatissime sono purtroppo ancora una tragica realtà. Lavoro nero sommerso che viene alla luce solamente nel momento della tragedia, dell'incidente che non può essere minimizzato o nascosto. E allora non siamo d'accordo con il ministro Sacconi: le regole e le sanzioni sono necessarie, altrimenti non si capisce come si possa richiamare le imprese alle proprie responsabilità. Il decreto correttivo approvato non ha fatto altro che abbassare livelli di tutela, deresponsabilizzare manager e dirigenti (che, invece, della sicurezza sono i primi responsabili), ridurre i poteri e le funzioni degli organismi di vigilanza, in totale dispregio di norme costituzionali e direttive europee. la vera urgenza di fronte alla strage continua nei luoghi di lavoro. Allargare le maglie della vigilanza, così come ha fatto il Governo, significa aver dato in sostanza il via libera al non rispetto delle più elementari norme che tutelano la vita dei lavoratori. È necessario rimuovere il blocco del *turnover* e integrare quelle 200 unità mancanti tra gli ispettori del lavoro dell'INPS, di cui parla il presidente Mastrapasqua nella sua audizione, affinché si possa intensificare l'attività di controllo. Noi vogliamo pene giuste e certe per i responsabili, ma anche sanzioni amministrative che sappiano colpire le imprese disoneste e salvaguardare quelle oneste e in regola, attraverso l'espulsione dalle associazioni di categoria, ma soprattutto, nei casi più gravi,

è arrivato il momento di aprire una discussione che riporti l'uomo, inteso come soggetto dotato di doveri, diritti e soprattutto dignità, al centro del processo produttivo. A questo dobbiamo cercare di arrivare, insieme, ognuno con il proprio ruolo: istituzioni, imprese, organizzazioni sindacali. Occorre ripristinare una cultura della sicurezza nei lavoratori e nei dirigenti, in grado, se necessario, di andare oltre la cultura del profitto. Occorre mettere le imprese di fronte alla loro cosiddetta responsabilità sociale, diffondendo lo sviluppo dell'etica imprenditoriale ed aiutandole attraverso politiche di formazione ed informazione, indispensabili per la prevenzione degli incidenti e la tutela dei lavoratori. Alla Commissione riconosciamo di aver svolto una meritoria indagine conoscitiva sull'argomento, ma auspichiamo che adesso si passi ad una seconda fase, in cui la Commissione rafforzi la sua istruttoria, anche con un più alto numero di missioni sul campo, e quindi formuli precise proposte che possano dare vita a leggi il più possibile condivise, scevre da pregiudizi di parte, migliorative dell'attuale testo unico, che riteniamo insufficiente per fronteggiare un fenomeno di tale portata. Più sarà completa, a 360 gradi, l'attività della Commissione, più incisiva potrà essere la normativa che scaturirà dai suoi lavori. È per questo che abbiamo ritenuto necessario presentare una nostra risoluzione, che impegni il Governo su alcuni punti che riteniamo imprescindibili. Chiediamo che il Governo si impegni a dare piena attuazione del decreto n. 81 del 2008 e ne ripristini l'impianto sanzionatorio successivamente modificato dal decreto correttivo n. 106 del 2009; che si adoperi affinché tutti gli organismi coinvolti, a partire dal Ministero del lavoro, forniscano, con tutti gli strumenti a disposizione, una puntuale informazione sulla normativa vigente, anche per fare in modo che tutte le parti in causa dispongano di una interpretazione certa e di una applicazione uniforme delle disposizioni; che vengano destinate risorse economiche ed umane congrue affinché gli enti preposti ai controlli e alla repressione di eventuali violazioni possano esercitare pienamente le loro funzioni; che si rafforzi il coordinamento e la collaborazione tra tutti gli enti istituzionali che si occupano a vario titolo della salute e della sicurezza sul lavoro, nell'intento di offrire alle imprese e ai lavoratori un approccio univoco e coerente della pubblica amministrazione sia nell'interpretazione delle norme che nella loro applicazione; che si assumano iniziative legislative rispettose delle disposizioni comunitarie, tese ad evitare che il principio del massimo ribasso d'asta sia considerato l'unico determinante di selezione delle offerte nelle gare d'appalto; si favorisca lo sviluppo della cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, sia attraverso corsi nelle scuole sia con la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro, con particolare attenzione alle piccole e medie imprese. Infine, chiediamo di rivedere la normativa in materia di assicurazione contro gli infortuni domestici, ampliando il più possibile la tipologia dei sinistri coperti dall'assicurazione e abbassando la soglia di inabilità necessaria per usufruire dell'indennizzo,

la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro si è occupata sin dall'inizio della XVI legislatura di incidenti in ambito domestico istituendo un apposito gruppo di lavoro, acquisendo i dati necessari alla comprensione della reale situazione ed ascoltando i pareri e le analisi di tutti i soggetti coinvolti nella prevenzione e nella cura dell'infortunio in casa. La legge n. 433 del 1999 ha equiparato, almeno in linea di principio, il lavoro domestico a qualsiasi altra attività lavorativa, riconoscendo dunque pari dignità al lavoro di oltre cinque milioni di casalinghe. La legge ha poi istituito un sistema di raccolta dati presso l'Istituto superiore di sanità ed ha stabilito l'obbligo di assicurazione per la tutela del rischio infortunistico per invalidità permanente da lavoro svolto in ambito domestico, dando all'INAIL, ai Ministeri competenti e alle associazioni di categoria la responsabilità di gestire un fondo autonomo speciale che ha il compito di raccogliere i premi e pagare le rendite. A dieci anni dall'entrata in vigore della legge è stato necessario tracciare un bilancio: la legge n. 433 del 1999 non ha ridotto gli infortuni in ambito domestico, e l'assicurazione obbligatoria vive una situazione di stallo preoccupante. Risultati positivi sono riscontrabili solo nella raccolta dati e nell'analisi del fenomeno. In altre parole, adesso abbiamo un quadro più chiaro sugli infortuni domestici. i progressi tecnologici e le scoperte in campo scientifico hanno reso più sicure le cucine (dove avviene il 58 per cento degli incidenti che coinvolgono donne), gli impianti di riscaldamento e gli elettrodomestici, ma non hanno ridimensionato significativamente il fenomeno. Il numero dei morti a seguito di incidente in ambito domestico è ancora molto elevato. Il dato non è uniforme né oggettivo, in quanto ogni istituto di ricerca utilizza metodologie differenti di classificazione: secondo l'Istituto superiore di sanità i decessi sarebbero 5.500,

le donne tra i 18 e i 65 anni che muoiono ogni anno a seguito di incidenti in casa sono 450, mentre 900 circa restano invalide in modo permanente.

cento dei casi di soffocamento riguarda le donne, i casi di folgorazione riguardano donne per il 70 per cento e i casi di ustione riguardano donne per il 60 Esiste dunque una condizione di rischio assimilabile al rischio professionale presente in qualsiasi industria o fabbrica. L'esposizione a sostanze tossiche, così come l'utilizzo di apparecchi domestici, è un problema serio che espone la casalinga ad un rischio di breve termine, legato soprattutto all'uso di sostanze caustiche, ma anche ad un rischio a lungo termine ancora poco studiato. Il numero di decessi e infortuni in casa è dunque estremamente preoccupante nonostante il livello di allarme sociale sia molto basso. La percezione di casa come luogo sicuro aumenta inoltre il rischio di infortunio, se si considera che le principali cause di incidente sono la distrazione e l'inappropriatezza dei comportamenti, più che il malfunzionamento degli elettrodomestici o degli impianti a gas. Dai dati presentati emerge la necessità di concentrare gli sforzi del legislatore sulla prevenzione. Alcune Regioni, così come previsto dalla legge n.

ha tra i 18 e i 64 anni ed il 28 per cento ha più di 65 anni. Per le donne in età lavorativa, è stata studiata la possibilità di inserire nei corsi preparto alcuni incontri di formazione sugli infortuni domestici, mentre per la fascia di età più elevata gli strumenti predisposti appaiono scarsamente efficaci: in particolare, opuscoli informativi spesso complicati o pubblicazioni scientifiche *on line* pur se facilmente reperibili, *de facto* vengono consultate solo dagli addetti ai lavori. Per questa fascia di età bisogna passare attraverso i centri anziani presenti sul territorio e soprattutto attraverso la televisione nazionale e locale, che è in grado di veicolare il messaggio anche presso le persone che vivono in condizione di emarginazione e solitudine. In questo senso risulta incoraggiante, anche se ancora insufficiente, la mini *fiction* trasmessa durante il programma "Uno Mattina" della RAI sulla famiglia Sbadatelli, dove si spiega quali sono i comportamenti da evitare in casa. Le risorse per incrementare l'attività di prevenzione non mancano. Il Fondo speciale per gli infortuni in ambito domestico, istituito presso l'INAIL, ha un avanzo patrimoniale di circa 93.693.000 euro ed un avanzo economico 9.209.000 euro. Tale dato non può essere considerato meramente come positivo. L'erogazione di rendite si è infatti praticamente bloccata e le casalinghe continuano a pagare i premi assicurativi senza di fatto ricevere né il risarcimento in caso di infortunio né un'adeguata attività di prevenzione. Dal 1° marzo 2001 al 31 dicembre 2008 sono state presentate 10.920 domande delle quali 9.782 sono state definite negativamente e 692 si trovano in fase istruttoria, mentre sono solo 446 su 10.920 le rendite effettivamente erogate. Nei primi sei mesi del 2008, poi, sono state pagate solo 3 rendite (delle quali 2 riguardano incidenti mortali). L'assicurazione obbligatoria riguarda le persone in età compresa tra i 18 e i 65 anni che svolgono attività in ambito domestico per la cura del nucleo familiare e dell'abitazione e che non siano impegnate in altra attività lavorativa. Secondo l'ISTAT sono 5.200.000 le persone che rientrano in questa categoria, ma al 31 dicembre 2008 risultano iscritti solo circa 2.167.000 soggetti, dei quali 199.748 hanno un reddito complessivo lordo ai fini IRPEF inferiore a 4.648 euro (per i quali dunque l'iscrizione sarebbe gratuita). Essendo inoltre il premio già particolarmente basso (12,91 euro l'anno), i motivi per i quali la metà delle casalinghe non si assicura possono possono essere solo la scarsa conoscenza della norma o la scarsa fiducia nei confronti dell'INAIL, che rigetta l'87 per cento delle richieste di risarcimento o tiene da diversi anni ben 927 casi in istruttoria. A seguito delle audizioni dei rappresentanti di INAIL, ISPESL e ISS in Commissione infortuni è emerso il dato che il 65 per cento delle domande viene rigettato in in quanto l'invalidità cagionata da incidente domestico è al di sotto della soglia fissata per legge. L'abbassamento del grado minimo di indennizzabilità dal 33 al 27 per cento disposto dalla finanziaria del 2007 non è stato sufficiente ad aumentare considerevolmente il numero delle rendite pagate: solo 44 infortuni in più sono stati riconosciuti dall'INAIL nella soglia di danno compresa tra il 27 e il 33 per cento. Appare dunque evidente che l'assicurazione contro gli infortuni domestici è, ad oggi, un fallimento e che l'unico modo per convincere le casalinghe a versare il premio ed obbligare l'INAIL a pagare le rendite è abbassare la soglia dell'indennizzo avvicinandola a quella degli altri lavoratori. Un eventuale aumento del pagamento delle rendite non porterebbe automaticamente alla diminuzione dell'avanzo di 9.209.863 euro, in quanto ad oggi solo il 50 per cento delle casalinghe paga il premio assicurativo. Rendendo il sistema più trasparente ed efficiente l'aumento dei versamenti da parte delle casalinghe potrebbe compensare l'aumento del pagamento delle rendite, rendendo ancora disponibili sufficienti risorse per un programma di prevenzione nazionale concentrato sulle televisioni nazionali e locali. *(Applausi dal Gruppo PdL. Signora Presidente, signor Sottosegretario, colleghe e colleghi, la frequenza del numero degli infortuni e delle morti sul lavoro è una tragedia del nostro tempo alla quale si deve e si può reagire. Non possiamo rassegnarci alla drammatica cadenza di una media di tre morti al giorno. Le malattie e gli infortuni, le condizioni di lavoro e le ricadute sulla salute ci segnalano una situazione rispetto alla quale l'attenzione e il controllo sono ancora del tutto insufficienti, mentre crescono i soggetti ed i lavori potenzialmente esposti a conseguenze pesanti rispetto alla propria salute ed integrità psicofisica. La crisi in atto spinge le imprese a comprimere i costi quanto più possibile ai fini della loro sopravvivenza ed è prevedibile che le prime tutele a cadere siano quelle legate alla sicurezza ed alla tutela della salute nei luoghi di lavoro. Lavoratori ed imprenditori, soprattutto nella piccola e media impresa e nelle aziende artigiane, sono accomunati nell'accettare implicitamente l'innalzamento delle soglie di rischio pur di difendere la sopravvivenza dell'impresa e del proprio lavoro, con le conseguenze drammatiche che poi ne conseguono al minimo errore umano o al mancato funzionamento di qualche protezione. Alle vecchie emergenze se ne aggiungono di nuove. Ed è per questo che è stato importante nel corso del Governo Prodi portare a compimento, con l'approvazione della legge n. 81 del 2008, il complesso e lungo processo legislativo in materia di salute e sicurezza, delineando un sistema complessivo consolidato, stabile e per la prima volta caratterizzato da una organica sistematicità; un *iter* legislativo mediante il quale si è portato a compimento un impegno lungo oltre trent'anni e che ha consentito di dare corpo ad un testo che raccogliesse, razionalizzandolo ed aggiornandolo, lo stratificato quadro legislativo in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Ironia della sorte: un compito così ambizioso lo ha raggiunto, nell'aprile del 2008, un Governo che non è riuscito ad arrivare al suo termine naturale. Il Governo attuale, sin da subito, non si è mosso nella direzione di dare immediata attuazione al quadro legislativo che ereditava, ma ha invece introdotto rinvii, proroghe, deroghe e modifiche che ne hanno rallentato l'entrata in vigore, nonostante la sicurezza sul lavoro resti una delle emergenze nella situazione lavorativa. Le modifiche perseguite in maniera pregiudiziale dal Governo ed introdotte con il decreto legislativo n. 106 del 2009 non hanno però modificato sostanzialmente i pilastri del decreto legislativo n. 81: primo, il campo di applicazione che prevede l'inclusione del lavoro autonomo e delle imprese familiari e di tutte le tipologie flessibili; il sistema istituzionale che definisce i livelli di coordinamento nazionale e periferico, il sistema informativo e le funzioni degli enti preposti; terzo, le misure generali di tutela e valutazione dei rischi con il documento di valutazione dei rischi che include l'organizzazione del lavoro ed abolisce l'autocertificazione; gli obblighi connessi agli appalti, che ampliano la responsabilità solidale dell'appaltante; quinto, il sistema di rappresentanza basato sulla figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale e territoriale; infine, le misure a sostegno delle piccole e medie imprese.

Ora è necessario che il Governo ne acceleri la piena attuazione; su questo si dovrà concentrare il lavoro di stimolo della Commissione, ed il lavoro svolto in questi mesi ci consente di focalizzare con maggiore chiarezza gli ambiti sui quali incentrare l'azione del legislatore. La crisi, come già ho detto prima, porta alla sottovalutazione dei pericoli ed all'innalzamento delle soglie di rischio. Le malattie professionali sono un tema ancora poco approfondito l'evoluzione dell'organizzazione del lavoro non è accompagnata da informazioni utili a comprendere ed a conoscere la pericolosità di sostanze, strumentazioni e condizioni di lavoro che possono pregiudicare nel tempo e stabilmente le condizioni psichiche e fisiche delle lavoratrici e dei lavoratori. Il lavoro irregolare è in aumento, e segnali molto precisi ci indicano che il lavoro minorile non è un fenomeno dei Paesi poveri, ma è presente nel nostro Paese e colpisce soprattutto le fasce più povere ed emarginate. La salute oggi non è considerata dal Governo non è considerata dal Governo come una priorità: a partire da quella sul piano generale è oggetto di tagli sempre più consistenti. Con questo esempio come potrebbe essere quella nei luoghi di lavoro? Le soglie di rischio si stanno innalzando a livelli inaccettabili. Sono scomparse le rilevazioni sulle ricadute psichiche in termini di benessere generale. Si è abbassata l'attenzione ed è calato il silenzio sugli aborti bianchi nel mentre si ideologizza la RU-486. I luoghi e gli ambienti di lavoro sono l'ultimo degli interventi ispettivi, visto che visto che gli ultimi potenziamenti di organico sono stati quelli fatti dal ministro Damiano. C'è molto lavoro per la Commissione, ma dobbiamo rendere più efficace il ruolo che stiamo svolgendo con una più puntuale presenza, non solo in occasione di eventi tragici e significativi, ma soprattutto allargando l'azione a tutte le attività di indagine che alla Commissione sono state assegnate, con risorse adeguate e in grado di consentire di far fronte a questi impegni. Molte indicazioni sono venute nel corso delle numerose audizioni svolte, e la relazione che stiamo discutendo ne dà ampio riscontro. Raccogliendo le numerose sollecitazioni, venute in particolare dal Presidente della Repubblica nel corso di questi anni, dobbiamo aumentare ancor di più l'impegno e non adagiarci sui segnali di inversione di tendenza che ultimamente si sono registrati, così da dare al nostro Paese la speranza che di lavoro non si sia condannati a morire.

la Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni sul lavoro è stata istituita dal Senato praticamente in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto ed ha avviato i lavori contestualmente all'elaborazione e all'emanazione dello schema di decreto legislativo correttivo ed integrativo del 2 agosto 2009, Il decreto n. 81 fu emanato - è bene ricordarlo - a Camere praticamente sciolte ed in maniera un po' frettolosa, sull'onda emotiva di avvenimenti luttuosi che avevano inevitabilmente spinto ad enfatizzare profili più propriamente sanzionatori della nuova disciplina, tanto da far definire lo stesso, non solo dal mondo datoriale ma anche da tanti studiosi, come inutilmente punitivo e repressivo. Ciò che a tanti apparve certo fin da allora - senza per questo disconoscere la validità, l'utilità e la necessità di un intervento teso al coordinamento della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di lavoro - fu la fretta con cui fu emanato, fretta che, fra l'altro, diede luogo ad un decreto che comprendeva diverse ed inutili ripetizioni e più di un errore: errori non formali vorrei dire, che, tra l'altro, potevano incidere negativamente sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. Bene ha fatto quindi, secondo noi, l'attuale Governo ad emanare, utilizzando una possibilità prevista nella legge delega n. un decreto correttivo ed integrativo inserito comunque all'interno dei principi e dei criteri direttivi di delega di cui alla legge n. 123, che qualcuno ha già battezzato come seconda riforma, proprio in ragione della portata delle novità introdotte. Come è intuibile, la Commissione monocamerale sulle morti bianche è stata in questi mesi impegnata sul decreto legislativo n. 81 e, ancora di più, sullo schema di decreto correttivo n. 106, approvato dal Consiglio dei ministri nell'agosto 2009. A tal proposito appare opportuno ricordare - lo ha già detto il presidente Tofani - quanto rilevante sia stato in particolare il contributo apportato dalla Commissione sulle morti bianche relativamente alla discussione degli articoli 2-*bis* (presunzione di conformità) e 10-*bis* (obbligo di impedimento), con l'emanazione peraltro di un proprio parere sugli articoli sopra citati, che lasciavano intravedere profili di incostituzionalità e che apparvero a molti come una riduzione dei livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Colgo l'occasione per esprimere il mio personale apprezzamento per l'atteggiamento del Governo e, per esso, del ministro Sacconi il quale - consentitemelo - da vero riformista si è reso disponibile a modifiche sostanziali dell'impostazione originale del decreto che aveva registrato, oltre ad un parere negativo espresso dalle Regioni e Province autonome, anche numerosi rilievi avanzati dalle Commissioni lavoro di Camera e Senato. La stesura definitiva del decreto legislativo n.

anche se persiste, e non potrebbe essere diversamente, qualche perplessità. Siamo tutti consapevoli, infatti, che le questioni che ci sono davanti sono riconducibili ad un tessuto normativo dinamico, che richiede una periodica manutenzione ed un continuo aggiornamento, imposte peraltro dalla continua e tumultuosa evoluzione tecnologica e dal processo di innalzamento della cultura sociale in materia di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro. In tale direzione la Commissione sulle morti bianche sta tuttora indagando con l'obiettivo di affrontare progetti specifici su particolari settori del mondo infortunistico che, anche perché poco o affatto indagati, si manifestano piuttosto complessi. Ma su alcuni di questi aspetti tornerò successivamente. L'esperienza vissuta intorno allo schema di decreto legislativo proposto dal Governo è stata quindi positiva sia per ciò che attiene i rapporti Governo-Parlamento sia per ciò che attiene i rapporti Stato-Regioni. testimonia ancora una volta, se mai ve ne fosse bisogno, che un confronto corretto fra Parlamento e Governo e tra Governo e Regioni, per tutto quanto è materia concorrente, è sempre possibile ed utile, anche perché il confronto consente di raggiungere più elevati risultati che, nel caso in argomento, sono fondamentali in quanto riguardano il bene primario della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. Ed è in questo spirito, quello cioè del confronto franco e proficuo tra Governo e Parlamento e fra Stato e Regioni, nel segno di un federalismo positivo, che vorrei continuare il mio intervento sviluppando alcune ulteriori riflessioni circa il decreto A parere di chi parla il Governo dovrebbe perseguire con maggiore fermezza e con rinnovata tenacia, anche attraverso i decreti e le norme attuative, nello spirito della più ampia condivisione e partecipazione sociale, i seguenti obiettivi: sviluppo di una maggiore integrazione tra gli attori della sicurezza sui posti di lavoro (i lavoratori ai diversi livelli di responsabilità), anche promuovendo azioni operative in stretta sinergia che coinvolgono i principali soggetti interessati al sistema prevenzionistico; promozione e l'armonizzazione degli interventi di vigilanza e di controllo degli enti istituzionalmente preposti, impegnando di conseguenza più razionalmente risorse e professionalità.

del 2009 hanno avuto abbastanza coraggio per dar corso ad un superamento del sistema duale in materia di vigilanza e controllo; possibilità - vorrei ricordare - prevista dai criteri della legge delega. Speriamo che il Governo sappia rimediare alle criticità proprie di un sistema duale, vale a dire sovrapposizioni, duplicazioni e carenze, con le norme attuative; rimedio funzionale, tra l'altro, alla piena applicabilità di alcune norme del decreto legislativo n. 106 del 2009. Si pensi, ad esempio, alla difficoltà, in un sistema di vigilanza e controllo affidato a più soggetti e in assenza di una banca nazionale delle violazioni,

Inoltre occorrerebbe: rinforzare la pianificazione e l'implementazione di strategie d'intervento che, in stretta correlazione con le specificità produttive tipiche del territorio, tengano conto anche degli orientamenti delle istituzioni regionali; la previsione e la realizzazione di un centro informativo sulla tematica infortunistica e sulla casistica incidentale relativa ai mancati infortuni, quale banca dati per un confronto aggiornato e pertinente sulla natura e dimensione del fenomeno a livello nazionale e comunitario; lo sviluppo di un adeguato sistema di comunicazione in merito all'accesso a nuove forme di supporto economico e finanziario per le aziende, semplificando le procedure di accesso ed introducendo strumenti in grado di misurare l'efficacia nel tempo degli interventi effettuati; la promozione di azioni utili a favorire un maggior coinvolgimento ed un più partecipato consenso dei destinatari del procedimento normativo, con l'obiettivo della realizzazione di un ambiente di lavoro più confortevole e sicuro; la promozione, anche attraverso accordi sindacali, di codici etici di condotta quali punti di riferimento e di orientamento per i comportamenti di tutti gli attori presenti a vario titolo nella realtà aziendale; l'incentivazione all'adozione di modelli organizzativi, favorendone un'applicazione dimensionata sulle caratteristiche aziendali e sulle specifiche tipologie produttive. quindi individuati modelli di riferimento che, successivamente alla fase di prima applicazione della norma, possano coerentemente indirizzare gli interessati verso un idoneo e semplificato processo applicativo. L'adozione di tale modello risulterebbe quindi sempre necessaria, anche se il legislatore ha previsto la non sanzionabilità per la mancata applicazione. Occorre inoltre l'implementazione di azioni d'informazione e di formazione, in particolare verso i lavoratori stranieri, coinvolgendo anche il sistema territoriale della formazione ed istruzione (Province, scuole, università) nonché la realizzazione di matrici standardizzate per i modelli di valutazione del rischio lavorativo. Tale aspetto riveste particolare importanza al fine di normalizzare il metodo di redazione del Documento di valutazione del rischio (DVR) che costituisce l'elemento portante di tutto il sistema prevenzionistico inserito nei contenuti del Il Documento costituisce, di fatto, non solo lo strumento di valutazione dei rischio lavorativo, ma anche il mezzo per l'indicazione delle relative misure di prevenzione e protezione necessarie alla riduzione ed all'eliminazione dei rischi mansionali. In tal senso appare necessario predisporre nei decreti e nei regolamenti attuativi un modello dinamico di Documento di valutazione del rischio, con relativo schema ed applicabile alle specificità aziendali e produttive maggiormente rappresentative del Paese. l'avvio di ulteriori azioni utili a garantire il governo di tutto il processo di informazione, formazione e addestramento del personale sulla prevenzione dei rischi lavorativi, operando con adeguate progettazioni ed in conformità al contesto produttivo interessato (tali iniziative dovranno essere realizzate secondo specifici sistemi di qualità), dei contenuti previsti dal sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi anche a tutte le altre tipologie produttive, al fine di realizzare la cosiddetta «patente a punti dell'azienda» che sempre più dovrebbe costituire elemento di riferimento obbligatorio (e non solo preferenziale) per la partecipazione alle gare di appalto, subappalto, accesso a contributi, finanziamenti, agevolazioni. Occorre ribadire la centralità dello Stato sulla normalizzazione dei sistemi e metodologie di controllo della salute e sicurezza sul lavoro, anche come soggetto promotore di azioni tese ad implementare la cultura della salute e della sicurezza sul lavoro, elemento che può rappresentare un valido misuratore del grado di civiltà di un Paese. Un contributo importante può venire, in tal senso, dalla Commissione parlamentare di inchiesta sugli infortuni e sulle morti bianche che, si è detto, ha come obiettivo la produzione di progetti e proposte solutive in merito a tali problematiche. A tal proposito, il lavoro della Commissione, come è stato ribadito anche dal Presidente, è stato organizzato

Al sottoscritto è toccato il ruolo di coordinare il gruppo di lavoro destinato ad indagare sugli infortuni *in itinere* e sulla complessità degli infortuni legati al settore dei trasporti. Ai colleghi vorrei ricordare che il comparto dei trasporti è uno dei più importanti settori produttivi del nostro Paese: esso presenta oltre 1.142.000 addetti e circa 166.000 società operative. Si tratta di un settore che, purtroppo, ha visto in questi anni una crescita incrementale anche sul versante degli infortuni lavorativi, con gravi perdite umane ed elevati costi economici per i lavoratori e per le aziende. In particolare gli incidenti stradali costituiscono ormai in Italia, come nel resto d'Europa, una vera e propria emergenza sociale e sanitaria. La Commissione ha avvertito, quindi, la necessità di elaborare uno specifico progetto sulla sicurezza dei trasporti che, da una parte, studi la dimensione reale del problema infortunistico ed individui i settori che espongono maggiormente a tale rischi i lavoratori per frequenza e gravità; dall'altra, indichi una scala di priorità per settore di appartenenza (stradale, ferroviario, aereo, marittimo) ed elabori una serie di azioni e di indirizzi di carattere tecnico, procedurale, organizzativo e normativo per contenere e abbattere tale fenomeno. Lo scopo dell'intervento è prevedere la prevenzione degli infortuni sul lavoro derivanti da incidenti in orario di lavoro e *in itinere* a partire da quelli che interessano il settore stradale; proporre, attraverso interventi ed azioni, l'attuazione e l'articolazione delle operazioni di verifica e controllo della sicurezza nella conduzione dei mezzi di trasporto e nelle verifiche costruttive e manutentive dei mezzi stessi; verificare le attitudini personali e le specifiche attività mansionali degli addetti attraverso un sistema di gestione dinamico in grado di favorire l'ottimizzazione delle attuali risorse e dei mezzi di lavoro impiegati sul territorio; coinvolgere enti e soggetti esterni professionalmente competenti in grado di valutare tutti i parametri necessari alla migliore tutela della salute e sicurezza, non solo del ma anche degli altri soggetti su cui potrebbero ricadere gli effetti di azioni scorrette o omissioni nel campo della sicurezza. In ultima analisi, lo scopo di tale proposta-progetto può essere sintetizzato nella promozione di una serie di azioni tese a realizzare la certificazione di un processo e di linee guida di indirizzo nell'ambito della sicurezza dei trasporti, realizzando un sistema prevenzionistico dei trasporti (un SPT)

destinate a modificare atteggiamenti non conformi alle norme e abitudini anomale che rappresentano, in percentuale, uno degli elementi di maggior causa del fenomeno infortunistico Molti sono gli argomenti che meritano sicuramente approfondimenti e impegno per la ricerca di soluzioni adeguate e su cui andrà sollecitata l'attenzione e l'azione del Governo. Basti evidenziare, ad esempio, come vi sia sperequazione di responsabilità applicativa a carico del datore di lavoro di un'azienda quando, in occasione di un evento infortunistico *in itinere* (e quindi senza alcuna responsabilità dello stesso in merito alle cause dell'evento),

l'intera problematica relativa agli infortuni sui luoghi di lavoro, con azioni che coinvolgano tutti gli attori e in particolare i lavoratori, non solo quali soggetti destinatari del sistema prevenzionistico di cui al decreto legislativo n.

siamo sicuri - un abbattimento progressivo nel tempo del fenomeno infortunistico che rappresenta, purtroppo, ancora oggi uno dei problemi più gravi del Paese in termini di perdita di vite umane e in termini economici. *(Applausi

Signora Presidente, mi unisco innanzitutto all'auspicio del presidente Tofani di continuare in un lavoro connotato da un forte spirito collaborativo e dalla volontà di aggredire uno dei problemi sociali più gravi del nostro tempo. Il punto focale della Relazione intermedia che oggi discutiamo è, a mio avviso,

i numeri però in Italia continuano ad essere altissimi e questo è inaccettabile in un Paese civile, come più volte, anche recentemente, ha affermato il presidente della Repubblica Napolitano.

dobbiamo però sapere che da questa tragica contabilità sono esclusi tutti i lavoratori morti per le strade, come gli autotrasportatori o gli addetti alla manutenzione stradale; diversamente i morti sarebbero 700.

promuovere provvedimenti di rottamazione anche per le macchine agricole.

Se certamente possiamo considerare che l'attenzione vigile e continuata delle massime istituzioni, compresa la Commissione d'inchiesta del Senato, ha di certo contribuito a creare una rinnovata sensibilità ed un clima di attenzione, ciò nonostante il permanere di una misura tanto rilevante di incidenti anche gravissimi e mortali indica innanzitutto come la crisi che stiamo vivendo possa modificare, in peggio, le condizioni del lavoro, e abbassare anche la sensibilità verso gli obiettivi e i vincoli di sicurezza e salute nel lavoro e del lavoro, sia dei lavoratori che degli imprenditori, tutti protesi a salvare comunque l'azienda. Nella crisi tutti i diritti si fanno ancora più fragili, in un panorama italiano che ha già visto franare complessivamente i diritti del lavoro. Diritti che appartengono ormai ad una porzione delle forze del lavoro dipendente che va via via sempre più a restringersi. La stessa riduzione e scarsità delle risorse, sia quelle pubbliche -pensiamo a tutto il comparto dei trasporti pubblici - che private disponibili vede, di fatto, un riorientamento delle risorse stesse a discapito della qualità, della prevenzione, della sicurezza, a cui vengono sottratti investimenti significativi. I gravi, gravissimi incidenti degli ultimi tempi, come quello di Viareggio, largamente annunciato, che ha seminato tanto orrore e che non si può considerare una tragica fatalità, ci dicono proprio questo: quando si abbassa l'asticella dell'attenzione e la sensibilità sociale verso la sicurezza

che rendono possibile la sicurezza) si abbassa anche la soglia della prevenzione e si mettono a rischio tante vite umane. Allora dobbiamo valutare con chiarezza il rischio che il nostro Paese esca dalla crisi in peggio, sia per quanto riguarda i valori - i gravi fatti di xenofobia e di razzismo ce lo dimostrano - sia per le condizioni di sicurezza e giustizia sociale, con più disoccupazione, più precariato e meno diritti. Le stesse parole pronunciate in più occasioni dal presidente Napolitano ci invitano a guardare la crisi come un'occasione per farne uscire un'Italia più giusta. Ciò significa un'Italia più attenta ai valori del lavoro, alle tutele del lavoro e ai diritti del lavoro,

tendenza a ricorrere più largamente al lavoro sommerso, all'estensione dell'area del precariato e del lavoro irregolare, e perché cresce e non si riduce il ricorso all'impiego illegale di immigrati, nonostante la recente legislazione. Non abbassare la guardia, dunque. Questo deve essere lo spirito della nostra azione politica e parlamentare. E in questo spirito dovremo monitorare in pratica gli effetti della normativa recentemente modificata. In tal senso, le modifiche apportate al Testo unico del cosiddetto decreto Sacconi hanno purtroppo veicolato un messaggio negativo proprio alle categorie più esposte: quello di una riduzione delle tutele, del potere di deterrenza delle norme, dell'abbassamento della responsabilità manageriale e delle misure di protezione e prevenzione. Tutto questo non è un bene, e spetta a tutti noi vigilare e correggere quelle norme che effettivamente dovessero produrre questi gravi risultati. Signora Presidente, nella seduta di oggi affrontiamo, come è del tutto evidente, un grave problema sociale. Come sottolineato nella Relazione intermedia sull'attività svolta dalla Commissione d'inchiesta, in Italia ogni anno continua a verificarsi un elevato numero di infortuni e di decessi sul lavoro. Nel corso del 2008 abbiamo registrato 1.100 incidenti mortali, 875.000 infortuni e 28.000 malattie professionali. Anche se nello scorso anno, così come nel 2007, abbiamo registrato un andamento decrescente (ma non è stato così per le malattie professionali che, invece, sono in costante aumento) rimane un fenomeno gravissimo, assolutamente inaccettabile per un Paese civile come l'Italia. Le cause di un così elevato numero di infortuni e di infortuni mortali sono precise. In primo luogo, il permanere di una condizione lavorativa contraddistinta da una diffusa evasione dalle più elementari norme di sicurezza. In secondo luogo, la mancata formazione e informazione ai lavoratori e alle lavoratrici rispetto ai rischi lavorativi presenti quotidianamente nei luoghi di lavoro. Con l'entrata in vigore del decreto correttivo n. 106 del 2009, varato recentemente dal Consiglio dei Ministri, si è profondamente modificata la legislazione in tema di salute e sicurezza così come prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2008 varato dal Governo Prodi - voglio ricordare al senatore Morra - perché vi era una condizione sociale di estrema emergenza, sottolineata anche dal presidente della Repubblica Napolitano, sulla quale bisognava intervenire - altro che fretta! mentre da parte dell'opposizione - lo ricordo - anche nel corso della precedente legislatura si tendeva a rinviare continuamente il provvedimento, minimizzando questa gravissima piaga sociale. Signora Presidente, credo invece

aspetti sostanziali e di rilevante importanza, come quelli che riguardavano la presunzione di conformità alle prescrizioni e soprattutto l'obbligo di impedimento dell'evento lesivo che, incidendo sul codice penale, esonerava da responsabilità il datore di lavoro e interveniva in maniera concreta sui processi in corso, come nel caso drammatico della Thyssen.

gravi, perché intervengono negativamente sul Testo unico. Soprattutto viene meno, con questo intervento, la funzione di deterrenza che deve avere un sistema sanzionatorio che voglia davvero reprimere i comportamenti illegali. Come sapete e come

nel caso del decreto n. 106 non sono state rispettate queste condizioni prioritarie. Dobbiamo solo che le imprese non intendano queste nuove norme varate dal Governo come una loro sostanziale deresponsabilizzazione, riducendo così i livelli di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Speriamo davvero

la condizione preliminare di tutte le attività lavorative e non invece un costo da eludere, come capita sovente oggi. Inoltre, una vera azione di prevenzione richiede, ancora alle aziende, un forte impegno contro il lavoro nero e contro il cosiddetto lavoro grigio che, come sappiamo, contribuiscono in maniera considerevole ad aumentare il rischio lavorativo.

nel corso del 2008 hanno aumentato del 18 per cento - una misura significativa - la loro attività di controllo Se è così, diventa oltremodo necessario che anche il Governo faccia la sua parte e non emani, come nel caso dell'atto a firma del del ministro Sacconi, delle circolari ambigue dove per i controlli si chiede un intervento qualitativo piuttosto che quantitativo. A mio modo di vedere,

nel corso di questa legislatura, tale Commissione può davvero, e in parte lo ha fatto, rivestire un ruolo importante per approfondire ulteriormente le cause di questa gravissima piaga piaga sociale e soprattutto, come ha fatto in diverse occasioni, indicare al Parlamento le misure e gli interventi necessari per combatterla.

finestra"). Colleghi, vi informo che stanno assistendo ai nostri lavori gli studenti dell'Istituto tecnico per il turismo «Marco Polo» di Firenze, ai quali diamo il benvenuto. Dichiaro chiusa la discussione. Avverto che sono state presentate le proposte di risoluzione n. 1, a firma del senatore Tofani, relatore, n. 2, a firma del senatore Nerozzi ed altri, e n. 3, a firma della senatrice Bugnano ed altri.

credo che il dibattito di questa mattina abbia sicuramente fatto emergere un denominatore comune, chiaro ed evidente:

agli infortuni e per la certezza di avere luoghi di lavoro salubri. Ho particolarmente apprezzato anche i riferimenti alle malattie professionali, che stanno diventando un problema molto complesso. Non mi riferisco solo - è stato ben detto e richiamato - a quelle tabellate, ma anche e soprattutto a quelle non tabellate.

che i danni alla sua salute sono determinati da quella particolare malattia. Abbiamo visto anche altre parti d'Europa dove ci si aspetta l'onda lunga del dramma dell'amianto, problema che sicuramente non ci sfugge e che conosciamo anche nella nostra Nazione. C'è, insomma, la necessità di una sempre maggiore attenzione ai luoghi di lavoro e ai fenomeni nei luoghi di lavoro, perché i fenomeni collaterali, che non sono stati citati nella mia relazione ma che sono stati oggetto di questo anno di lavoro e anche di talune riflessioni da parte dei colleghi intervenuti, riguardano il rapporto umano all'interno del luogo di lavoro.

In questo ramo del Parlamento furono presentate ben 11 proposte, ma alla fine non si arrivò ad un percorso conclusivo. Ciononostante, la problematica esiste e vive e, quindi, quando parliamo di salute e di qualità nei posti di lavoro dobbiamo allargare a 360 gradi il nostro raggio d'azione. La Commissione, anche per i gruppi di lavoro che ha sta dando risposte importanti, significative e sostanziali, anche in quei settori dove sembrerebbe che tutto va bene, mentre non è così.

Questo significa che il dibattito di oggi, l'impegno della Commissione, la volontà di approfondire sempre di più e meglio questo tema per dare risposte, non dico esaustive, ma quanto più necessarie

specifiche collocazioni politiche, che vanno rispettate, e quindi anche delle diverse sensibilità che sono emerse su taluni punti,

Presidente, credo innanzitutto di dover esprimere apprezzamento nei confronti del lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta. Questa prima Relazione intermedia sull'attività della stessa

i temi e le questioni, i problemi che abbiamo di fronte determinando anche alcune indicazioni - credo condivise - impegnative nei confronti del Governo.

È stato il tentativo di continuare un percorso, riprendendolo là dove si era determinata una difficoltà di convergenza tra le parti sociali

cioè quello della formazione, cercando di attivare i meccanismi e le risorse utili, in collaborazione con le Regioni, per capitalizzare al meglio possibile gli interventi previsti all'interno della legge n. Tra l'altro, segnalo il fatto che su questo versante c'è molto da fare sul terreno della rapidità e della qualità degli interventi,

da una parte accelerare rispetto alla concretizzazione della norma; dall'altra, lavorare per verificare se e come, attraverso una sorta di avviso comune, fosse possibile intervenire in sede di definitiva

dalle risoluzioni presentate, in merito all'intervento del Governo in tema di regime sanzionatorio: noi riteniamo che molto si debba fare sul terreno

sul terreno del regime sanzionatorio un punto di equilibrio, ma non in direzione della deresponsabilizzazione;

che la questione della sicurezza è stata affrontata con una diffusa responsabilità istituzionale. Ha fatto bene il presidente Tofani a citare, tra le altre cose, lo sprone, l'insegnamento e l'incitamento

non mi cimenterò nella dialettica a proposito della tendenza positiva o negativa in relazione agli andamenti statistici ed alle cifre, perché tutti abbiamo la consapevolezza che finché ci sarà anche un solo sul lavoro non vi sarà statistica che tenga ed avremo tutti il dovere di affrontare comunque, con attenzione, impegno e mobilitazione, il tema che abbiamo di fronte. Mi permetto allora, in coerenza ed in conseguenza di questa ultima riflessione, di

la mobilitazione e la passione civile, credo sarebbe buona cosa se il Senato riuscisse a trovare una convergenza

Credo che ognuno di noi ritenga Facebook uno strumento di contatto e di socializzazione estremamente importante.

Nel giro di poche ore la bacheca di Andrea Cevasco, che riportava giudizi positivi sul Presidente del Consiglio e sul suo Governo, è stata oscurata ed egli non è riuscito in nessuna maniera a riattivare il suo *account*,

Leggo soltanto la frase iniziale: «Con questo comunicato gli appartenenti al gruppo Facebook "Le Brigate Rosse" vogliono rispondere alle accuse rivolte da alcuni organi di stampa...».

relative al carcere di Rovigo e a quello di Venezia, carcere maschile e femminile, le quali riassumono tre dei problemi relativi alla sovrappopolazione dei nostri istituti. Nel caso di Rovigo, infatti, esiste l'identificazione di un luogo dove dovrebbe essere costruito un nuovo carcere. Sono stati fatti i bandi per la costruzione dello stesso, ma non si è più avuta notizia in relazione il carcere di Rovigo è stato considerato dismesso e, quindi, anche la manutenzione ordinaria dello stesso non avviene più e i detenuti vivono in condizioni pessime, condizioni che ho potuto constatare di persona visitandolo Per quanto riguarda il carcere di Venezia, si rilevano due tipi di problemi. Nella parte maschile esiste un'ala con quasi 40 e - ahinoi! - in base alla prassi italiana, possibili 80 posti letto che non sono messi a disposizione dell'istituto, perché devono essere terminati i lavori di ristrutturazione e assegnate alcune guardie, e nella parte femminile convivono 5 bambini con le loro madri. nel corso dell'audizione in Commissione diritti umani, aveva fatto sapere che tanto a Venezia quanto a Firenze si era ormai decisa, anzi portata a termine, la divisione relativa all'ospitalità data a detenuti con figli minori di tre anni. Ma né a Firenze né a Venezia tutto ciò è avvenuto. Dico questo perché - e concludo giorno prima la data del deposito di questa interrogazione, cioè il 15 settembre, ci era stato comunicato che durante l'estate il ministro Alfano avrebbe presentato il piano carceri. non sono state date risposte alle varie interrogazioni parlamentari a seguito delle visite ispettive che 160 colleghi hanno portato avanti in tutta Italia, ma non esiste neanche il piano carceri, e nel frattempo continuano ad aumentare, in virtù dell'immigrazione clandestina, gli ospiti nei nostri istituti di pena. **Sulla

la questione dell'ENI di Monterotondo. I 49 lavoratori erano stati salvati dall'accordo tra i sindacati e l'ENI, accordo promosso da noi parlamentari, e rispetto al quale il Governo aveva informazioni di tre mesi prima. La questione che pongo alla Presidenza (al di là del merito della singola interrogazione, dalle malattie rare alle condizioni di rischio nel turismo, alle questioni che riguardano le frequenze nel momento in cui il digitale sta già cambiando la situazione) fatte in questo modo, signora Presidente, le interrogazioni e le interpellanze servono o non hanno forse cambiato natura? L'interrogazione o l'interpellanza di fatto serve a noi per incidere direttamente sui soggetti dell'interrogazione e dell'interpellanza e chiedere quindi

si è parlato con il vice ministro Urso in maniera interessante - credo - della ricerca e della ricerca applicata delle aziende italiane), allora non possono divenire un elemento di dibattito invece che essere confinate al campionato di serie B delle interrogazioni?

Presidente, la informo che, in sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento del Senato, il Gruppo dell'Italia dei Valori intende far propri i seguenti disegni di legge, già presentati e sottoscritti dal prescritto numero di senatori del Gruppo: Atti Senato nn. 1194, 1214, 1212, 1217, 1284, 1312,

1542, 1551, 1586, 1587, 1618, 1626, 1632,

un fatto molto grave, che riguarda i rapporti tra monopolisti, o ex monopolisti, come l'Enel, con i consumatori, gli utenti, le famiglie, soprattutto in una fase di crisi economica come l'attuale

durante le stagioni fredde come questa tolgano il servizio, secondo noi dell'Italia dei Valori è un atto di prepotenza, di arroganza e anche di illegalità, che contrasta con moltissime sentenze consolidate e con una giurisprudenza che fa prevalere il diritto alla salute rispetto agli interessi economici. Non è accaduto solo a Napoli,

in maniera brutale ed illegale ha staccato il riscaldamento ad un intero condominio, senza distinguere gli inquilini morosi da quelli in regola con i pagamenti, con grave danno all'integrità fisica di bambini, anziani e ammalati.

esistono i diritti di queste aziende a incassare le bollette, ma ci sono anche diritti alla salute che devono prevalere. Quindi, mi auguro che

con posizioni molto forti, che tranquillamente continuano ad operare, mentre altri, che cercano di avere contatti con altre persone per portare avanti ragionamenti politici - e non solo - vengono cancellati.